paradossale. Il gruppo Engineering, infatti, vanta 6.000 dipendenti e ha peraltro raggiunto nella difficile congiuntura del 2009 risultati fortemente positivi, con un utile netto di 34,3 milioni di euro, facendo registrare un balzo rispetto all'anno precedente del 131 il consiglio d'amministrazione ha deliberato la distribuzione di un dividendo di 0,565 euro per ogni azione. L'utile di esercizio del 2009 di Engineering.it è pari a 10,202 milioni di euro, più del doppio rispetto a quello 2008. Ecco perché,

stante questa situazione aziendale più che positiva, si ritiene necessario che siano poste in essere da parte dei responsabili del Gruppo Engineering tutte le azioni utili per una ricollocazione in azienda dei lavoratori collocati in anche in considerazione del recente decreto governativo che consente l'applicazione dei lavoratori in CIGS presso la propria azienda per processi formativi abbinati all'impiego lavorativo e come proposto dalle stesse organizzazioni sindacali dei metalmeccanici in un recente confronto Governo, noi chiediamo di sapere se il Ministero abbia un indirizzo e se intenda intervenire per risolvere una situazione veramente particolare e, ripeto, paradossale, proponendo eventualmente un altro incontro con il Ministro per riassorbire questi lavoratori.

il senatore Fosson nel presente atto parlamentare sollecita l'attenzione sulla situazione occupazionale della società Engineering spa, interessata da un processo di riorganizzazione con concessione di trattamento di CIGS. In proposito, informo il senatore che il giorno successivo alla pubblicazione del presente atto parlamentare, il 13 maggio scorso, si è svolto un incontro presso il Ministero del lavoro per la verifica della situazione aziendale, in attuazione dell'accordo del dicembre 2008. In quella sede, la società in parola ha illustrato l'andamento del piano di riorganizzazione dichiarando di aver adempiuto a tutti gli impegni previsti. In particolare, la società ha evidenziato che l'applicazione degli strumenti concordati per il riequilibrio degli organici ha consentito un andamento decrescente dell'utilizzo della CIGS; è stata, inoltre, confermata l'effettuazione dei corsi di formazione, previsti e illustrati nel precedente incontro di verifica, per il personale collocato in cassa integrazione straordinaria. Le parti hanno riconosciuto, come evidenziato anche nell'atto ispettivo, che il piano di riorganizzazione, in applicazione degli interventi preventivati, ha prodotto risultati positivi in termini di competitività e di riposizionamento sul mercato. Nel corso dell'incontro le organizzazioni sindacali hanno richiesto, ai sensi del decreto-legge n. 78 del 2009, l'utilizzo dei lavoratori in cassa integrazione in progetti di formazione o riqualificazione, che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento; ciò al fine di creare ulteriori opportunità di riassorbimento del personale sospeso. Al riguardo, però, la società, pur confermando la prosecuzione delle azioni previste per il reinserimento del personale sospeso, ha ritenuto che, al momento, il predetto strumento non offra utilità concrete in quanto i lavoratori potranno essere impiegati al termine del periodo di sospensione. A fronte di una siffatta situazione, cioè di una determinazione imprenditoriale

non ha potuto che prendere atto degli esiti della verifica in conformità del ruolo di mediazione e di conciliazione attribuito al Ministero stesso nell'ambito delle politiche occupazionali.

rimane sempre il fatto che comunque il Governo non è riuscito, di fronte ad una decisione imprenditoriale di questo tipo (mi permetta di dire paradossale), a far rientrare il paradosso di un'azienda che comunque lavora anche con lo Stato,

sottolineo quanto lei ha detto: credo nella possibilità di un nuovo incontro con l'azienda, con la mediazione del Governo; mediazione che chiedo sia anche più pesante per far eliminare o comunque

è stata introdotta con decreto ministeriale del 15 aprile 1994 senza la necessaria copertura finanziaria. A conclusione dei corsi i giovani conseguono, previo superamento degli esami di Stato, il diploma di istruzione professionale e, previo superamento degli esami regionali, la qualifica professionale di secondo livello nel quadro di specifiche intese sottoscritte tra i competenti uffici scolastici regionali e le singole Regioni. L'attuazione di detto decreto è stata accompagnata, sin dal momento della sua prima applicazione, da notevoli tensioni con il sistema delle Regioni per la mancata previa concertazione istituzionale. Ciò ha comportato che gli istituti professionali realizzano, nella maggior parte dei casi, soltanto i corsi surrogatori previsti dall'articolo 5 del medesimo decreto, in assenza di intese regionali, senza poter rilasciare attestati di qualifica riconosciuti dalle Regioni. Nell'anno scolastico 2008-2009 sono stati attivati in totale n. 8.023 corsi nelle quarte e quinte classi dei predetti istituti, di cui 4.571 corsi surrogatori, pari al 57 cento, e 3.452 corsi regionali pari al 43,6 per cento, che sono stati frequentati in totale da 140.409 studenti, di cui 60.065 iscritti ai corsi regionali e 80.344 iscritti ai corsi surrogatori. Sulla base degli esiti del monitoraggio effettuato periodicamente dall'Agenzia per lo sviluppo dell'autonomia scolastica è stata rilevata anche la estrema disomogeneità dei corsi di terza area attivati, in termini di numero di ore e obiettivi formativi. Per quanto riguarda il funzionamento della terza area, la mancata previsione nel bilancio di questo Ministero, sin dal 1995, di stanziamenti ordinari per il suo funzionamento, ha determinato una situazione di insostenibilità, che si è notevolmente aggravata per la diminuita disponibilità di risorse per le spese di funzionamento. Anche allo scopo di evitare che il problema finanziario si aggravi per l'ulteriore diminuzione delle risorse disponibili e che gli istituti professionali continuino a realizzare i corsi di terza area a carattere surrogatorio, i nuovi ordinamenti degli istituti professionali, che entreranno in vigore a partire dalle prime classi funzionanti nell'anno scolastico 2010-2011, hanno previsto la loro sostituzione con complessive 132 ore di attività in alternanza scuola-lavoro nelle quarte e quinte classi funzionanti, fino alla messa a regime del nuovo ordinamento dell'istruzione professionale. Faccio comunque presente che la direttiva ministeriale n. 93 del 30 aprile 2009, riguardante l'utilizzazione delle disponibilità finanziarie relative al Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui alla legge n. 440 del 1997, ha previsto la disponibilità, per l'anno 2009, di 30 milioni di euro per la realizzazione dell'alternanza scuola-lavoro, con particolare riferimento all'area di professionalizzazione degli istituti professionali.

le ore di alternanza scuola-lavoro che sono assolutamente indispensabili ed efficaci anche ai fini formativi della loro crescita scolastica e professionale.

una posta finanziaria che permetteva l'espletamento di questo monte ore e di questi *stage*; oppure il buonsenso e soprattutto il rispetto per la scuola viva e militante e per gli interessi collettivi

Mi pare assolutamente inutile prendere a pretesto il fatto che non ci siano state risorse finanziarie dal 1994 e che ci sia stata tutta una serie di condizionamenti dal punto di vista dell'economia, con riguardo in particolare al settore della scuola. Sul settore della scuola si è abbattuto di tutto: abbattuto di tutto: il taglio di 8 miliardi fatto nella finanziaria e tagli continui, che riguardano non soltanto il personale ma soprattutto la qualità perché quando si interviene tagliando le risorse naturalmente si incide pesantemente sulla qualità. Quale taglio peggiore sulla qualità

dell'*homo faber*. Abbiamo bisogno di gente professionalizzata, di gente che ha delle *performance* che possono essere immediatamente spese nel mondo del lavoro. Ebbene, tagliamo proprio i fondi che danno a questi giovani la

al pubblico, non è possibile tutto questo. Continuiamo a fare teoria, poi ci lamentiamo che dalle nostre scuola non vengono sfornati, così come si dice, ragazzi in grado di immettersi nel mondo del lavoro avendo già una capacità produttiva che interessi alle aziende e che pertanto li renda attrattivi. Se si continua a colpire la scuola in questo modo, se si continua a dire che non ci sono risorse per la qualità e per finanziamenti adeguati per questo tipo di istituti, che farebbero anche la qualità delle professioni nel mondo del lavoro (che oggi manca perché le aziende sono costrette a fare formazione per conto loro), la scuola non darà queste risposte. Di cosa parliamo? Di quale riforma? Coloro che avevano già iniziato un percorso avevano diritto a terminarlo: quando la partita è cominciata non si può intervenire per fermare un percorso cambiando le regole del gioco. Così ha fatto il Ministro e così continua a fare. Noi però non siamo soddisfatti e riteniamo che lo sciopero che i ragazzi hanno messo in atto

nel dettare disposizioni in materia di organizzazione scolastica, ha stabilito la sospensione delle procedure per l'accesso alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario attivate presso le università (SSIS) per l'anno accademico 2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti riguardanti la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso e la revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione degli organici del personale docente e ATA. Faccio presente inoltre che il decreto ministeriale n. 42 dell'8 aprile 2009, di integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2009-2010 e 2010-2011, prevede che possono presentare domanda di inserimento a pieno titolo nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento sia coloro che sono già in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso o per il posto cui aspirano, sia alcune categorie di aspiranti non ancora in possesso dell'abilitazione, tra i quali coloro che hanno frequentato i corsi del IX presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, che hanno conseguito detta abilitazione entro il 30 giugno 2009 e che hanno provveduto ad inviare la dichiarazione sostitutiva della certificazione concernente l'avvenuto conseguimento del titolo entro il medesimo termine del 30 giugno 2009. Anche coloro che hanno frequentato i corsi SSIS che si sono conclusi nella sessione autunnale del 2009 ed hanno chiesto di iscriversi nelle graduatorie ad esaurimento per il biennio 2009-2011 sono stati inseriti con riserva nelle graduatorie medesime. Infatti l'articolo 4, comma 6, del decreto ministeriale n. 42 dell'8 aprile 2009 prevede che «Coloro che per qualunque motivo non conseguono il titolo abilitante entro la data del 30 giugno 2009, ovvero non provvedono a inviare la citata dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno 2009, vengono inseriti con riserva in graduatoria. Con successivo decreto ministeriale sarà fissato il termine entro il quale sarà disposto lo scioglimento della riserva, previa autocertificazione del conseguimento del titolo, nei confronti dei docenti che conseguiranno l'abilitazione in tempo utile per le assunzioni relative all'anno scolastico 2010-2011». Con decreto n. 39 del 22 aprile 2010, è stato fissato per il 30 giugno 2010 il termine ultimo per gli adempimenti connessi allo scioglimento della riserva. Con nota del 10 marzo 2010, sono state fornite precisazioni, che non riguardano coloro che sono inseriti in graduatoria con riserva a seguito di ricorso giurisdizionale o al Capo dello Stato. Detto quanto sopra, per quanto concerne la richiesta di inserimento con riserva nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti iscritti per l'anno scolastico 2008-2009 ai corsi abilitanti COBASLID, AFAM di strumento musicale (classe 77/A) e scienze della formazione, preciso che tale possibilità non può essere concessa con un atto di carattere amministrativo, occorrendo una specifica norma di legge. Peraltro, in applicazione dell'articolo 2, comma 416, della legge del 24 dicembre 2007, n. 244, è stato predisposto lo schema di regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e della modalità della formazione iniziale del personale docente del sistema educativo di istruzione e formazione, che è stato inviato alle competenti Commissioni parlamentari per il prescritto parere. Al momento, risulta acquisito il parere delle Commissioni cultura e bilancio della Camera dei deputati.

far circolare la risposta che l'onorevole Sottosegretario ci ha fornito adesso fra tutte le persone che hanno cercato di prepararsi al meglio per garantirsi, con una professione sicura, anche una capacità qualitativa elevata. Chi fa i corsi di specializzazione lo fa perché vuole aggiungere qualità alla propria professionalità, ed è esattamente uno degli annunci uso la parola annunci, oramai, perché sarebbe stato invece un obiettivo acquisito da parte del Ministero quello della qualità e poi del riconoscimento del merito degli insegnanti, ma così non è. ma così non è. Onorevole Sottosegretario, la ringrazio perché, nel ricordare la data del 30 giugno 2010, ha avuto la cortesia istituzionale di rispondere oggi, che siamo ancora ancora lontani - si fa per dire - in termini burocratici dal 30 giugno 2010 e diamo la possibilità, con l'autocertificazione, di regolare la posizione a molti insegnanti. Ciò che turba ancora è la riserva, che deve essere sciolta dal Ministro dal momento che si trattava di un decreto ministeriale, il n. 42 dell'8 aprile 2009, e queste persone non possono vivere nell'ansia di non sapere. L'anno scolastico è incombente; siamo alla fine di un anno, ma anno, ma prima delle vacanze i dirigenti scolastici devono preordinare le classi. Arriverà un *annus horribilis*, onorevole Sottosegretario (lo annunciamo adesso, così quando accadrà nessuno si stupirà), perché avremo meno insegnanti in quanto, con le riforme della scuola secondaria di secondo grado ma anche di primo grado, sono state le classi disciplinari, ma non sono state modificate le classi di concorso, per cui abbiamo ancora delle graduatorie ad esaurimento che chissà quando si esauriranno. Allora, l'insoddisfazione mia

considerando che gli insegnanti sono un corpo femminilizzato - nella gran parte dei casi sono donne - con quello che ne deriva anche in termini sociali. Cosa voglio dire? Che vogliamo sollecitare il Governo; siamo in una sede appropriata, perché fra qualche giorno arriverà la manovra finanziaria. C'è una gran quantità di insegnanti che lascerà la scuola a causa del timore di perdere stipendio, aumenti di anzianità, TFR e pensioni.

Se rimane la riserva, rimane sospeso, sia per i dirigenti che devono fare le classi, sia per gli insegnanti che aspirano ad insegnare, il futuro. È una possibilità da non perdere per l'avvio di un anno scolastico che si annuncia comunque difficilissimo. Anche lei non ha potuto fare a meno di incominciare il suo intervento con la citazione dell'articolo 64 è il monumento alla distruzione della scuola. Quell'articolo ha già mandato fuori dalla scuola, nell'anno scolastico 2009-2010, 42.000 docenti e 15.000 personale tecnico e amministrativo. Nell'anno che incomincerà, oltre alla valanga di coloro che se ne vanno per paura di non poter contare su finanze certe e su redditi veri per la loro famiglia, avremo perciò l'uscita per raggiunti limiti di età e l'uscita

deve esaurirle. Dio non voglia che a causa anche di ciò che in quest'Aula e nell'altra Aula si aggira a seguito delle proposte della Lega - a cui questo Governo difficilmente dice di no - possano incominciare i concorsi regionali,

lunga e molto articolata. Nell'atto in discussione si afferma che per effetto delle misure previste dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 dalla legge n. 203 del 22 dicembre 2008 (legge finanziaria 2009) si è determinata una forte penalizzazione del Fondo per le supplenze conferite dai dirigenti scolastici, nonché del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche. Si afferma, inoltre, che si sarebbe determinata la penalizzazione del tempo pieno, facendo specifico riferimento alle scuole primarie di Milano e provincia. In primo luogo, vorrei ricordare che, come risulta dal Quaderno bianco sulla scuola presentato nel settembre 2007 dal precedente Governo, già allora era avvertita l'esigenza di interventi di razionalizzazione e di riqualificazione della spesa in materia di istruzione. Ciò trova conferma nella legge finanziaria 2007 nella quale si prevedeva, all'articolo 1, che con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione dovevano essere adottati interventi concernenti la revisione, a decorrere dall'anno scolastico 2007-2008, dei criteri e dei parametri per la formazione delle classi, al fine di valorizzare la responsabilità dell'amministrazione e delle istituzioni scolastiche scolastiche individuando obiettivi da attribuire ai dirigenti responsabili, articolati per i diversi ordini e gradi di scuola e le diverse realtà territoriali in modo da incrementare il volume e il valore medio nazionale del rapporto alunni-classe dello 0,4 per cento. Si sarebbe dovuto poi procedere alla revisione dei criteri e parametri di riferimento ai fini della riduzione della dotazione organica del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ATA. Gli obiettivi fissati dalla legge finanziaria 2007 sono stati conseguiti soltanto in parte, con la conseguente applicazione della clausola di salvaguardia prevista dalla stessa legge dalla stessa legge al comma 621 che ha comportato, da un lato una rimodulazione negli anni successivi dei tagli previsti e non operati e, dall'altro un taglio lineare degli stanziamenti del Ministero dell'istruzione. Da parte nostra abbiamo preso l'impegno di tenere sotto controllo i conti pubblici eliminando sprechi ed inefficienze. Come confermato dalle indagini dell'OCSE, le scuole italiane spendono mediamente per ciascuno studente molto più degli altri Paesi dell'area OCSE, ma i rendimenti in termini di istruzione sono al di sotto della media. Bisogna quindi restituire al servizio scolastico efficienza ed efficacia ed elevarne la qualità per avvicinarlo agli standard internazionali ed europei. Al raggiungimento di questi obiettivi mirano i provvedimenti normativi promossi dal Governo ed approvati dal Parlamento. Le misure e i provvedimenti assunti - inserendosi nel più ampio contesto della riqualificazione della spesa pubblica, anche in relazione alla difficile congiuntura finanziaria ed economica internazionale - hanno inteso salvaguardare quanto più possibile il sistema scolastico. Contrariamente a quanto avvenuto in passato, gli interventi previsti rientrano nell'ambito del processo di riqualificazione del sistema scolastico italiano e mirano a realizzare il riordino complessivo del sistema attraverso la valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, il pieno coinvolgimento delle Regioni e delle autonomie locali, una nuova *governance* territoriale dell'istruzione-formazione ed un più appropriato ed efficace utilizzo delle risorse. In questa ottica, quindi, si pongono le disposizioni dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, in materia di organizzazione scolastica, convertito dalla citata legge n. 133 del 2008, il cui impianto complessivo è stato riconosciuto costituzionalmente legittimo con sentenza n. 200 del 24 giugno 2009 della Consulta, che ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità sollevate sul comma 3 e sul comma 4, lettere da Quanto ai finanziamenti per il funzionamento amministrativo-didattico delle istituzioni scolastiche, faccio presente che sia nell'anno 2008, che nell'anno 2009 gli stanziamenti specifici (265 milioni di euro) sono stati azzerati in applicazione della suddetta clausola di salvaguardia introdotta dalla legge finanziaria 2007 che, come già detto, ha previsto interventi compensativi a decremento degli stanziamenti dell'amministrazione scolastica, a garanzia del raggiungimento delle economie sulle spese di personale da realizzare in attuazione dei commi da 605 al 619 dell'articolo 1. In particolare, per l'esercizio finanziario 2009 sono intervenute variazioni di bilancio pari a 60 milioni di euro per tutte le istituzioni scolastiche nazionali. Tali risorse sono state distribuite alle scuole che presentavano maggiori esigenze finanziarie, tenendo anche conto dell'incremento della popolazione scolastica. Le risorse, assegnate secondo detti criteri, costituiscono un incremento straordinario rispetto a quello programmato ed assicurato a tutte le istituzioni scolastiche. Per l'anno nota n. 9537 del 14 dicembre 2009, sono state fornite indicazioni alle istituzioni scolastiche per la compilazione dei documenti contabili per la programmazione del 2010, tenendo conto delle risorse finanziarie attualmente disponibili sui capitoli di spesa concernenti il personale e il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali; ciò per consentire alle istituzioni scolastiche una programmazione certa con riferimento alla dotazione finanziaria comunicata. Ulteriori indicazioni operative sulla predisposizione del programma annuale 2010 sono state poi fornite con circolare del 22 febbraio 2010. Relativamente alla gestione della cassa, specifiche indicazioni sono state fornite con circolare dell'aprile scorso, nella quale, fra l'altro, si è data informazione che è in corso di svolgimento, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'*iter* previsto dalla legge finanziaria 2010 per l'assegnazione a questo Ministero dei fondi relativi alle spese per il personale con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e per l'esternalizzazione dei servizi di pulizia a mezzo di contratti di servizio con ditte impieganti personale ex lavoratore socialmente utile. Con riferimento alle assegnazioni per le supplenze brevi e saltuarie conferite dai dirigenti scolastici, è stata assicurata preliminarmente una risorsa complessiva annuale ad ogni istituzione scolastica determinata sulla base del decreto ministeriale n. 21 del 2007; le maggiori esigenze che saranno rappresentate dalle istituzioni scolastiche (previo controllo del fabbisogno segnalato) potranno essere soddisfatte in considerazione dell'esigenza di garantire il diritto all'istruzione. Ciò è stato ribadito anche nella circolare del 10 marzo scorso, nella quale è stato, fra l'altro, fatto presente che «le richieste di maggior finanziamento per le spese di supplenza breve che le istituzioni scolastiche debbono sostenere per consentire l'ordinato svolgimento delle lezioni e, quindi, garantire il diritto all'istruzione» sono monitorate mensilmente tramite i flussi finanziari che le medesime devono trasmettere al Sistema informativo dell'istruzione. In merito, poi, alla circolare ministeriale n. 37 del 13 aprile 2010 e alla rilevata circostanza che gli Uffici scolastici regionali stanno predisponendo le dotazioni organiche e la strutturazione delle classi sulla base dello schema di decreto interministeriale diffuso con la stessa circolare, nelle more del perfezionamento del decreto stesso, vorrei ricordare che la prassi amministrativa di anticipare con una circolare i contenuti dello schema di decreto sulle dotazioni organiche nazionali è stata seguita anche dalla precedente gestione per le note ed ineludibili esigenze di carattere organizzativo preordinate all'ordinato avvio dell'anno scolastico. Per quanto riguarda specificamente il tempo pieno nella scuola primaria, nella suddetta circolare n. 37 è stato precisato che nulla è innovato e che, pertanto, restano confermati l'orario di 40 ore settimanali per classe, comprensive del tempo dedicato alla mensa, l'assegnazione di due docenti per classe e l'obbligo dei rientri settimanali. È stato inoltre evidenziato che le 4 ore residuate rispetto alle 40 settimanali per classe (44 ore di docenza a fronte delle 40 di lezioni e di attività), comunque disponibili nell'organico di istituto, potranno essere utilizzate prioritariamente per l'ampliamento del tempo pieno sulla base delle richieste delle famiglie e, in subordine, per la realizzazione di altre attività volte a potenziare l'offerta formativa (compreso il tempo mensa per le classi che attualmente praticano i rientri pomeridiani). Ovviamente, il tempo pieno può essere attivato solo in presenza di strutture e servizi idonei. Tutto ciò premesso sul piano generale, vengo a quanto rappresentato nell'interrogazione circa la paventata mancata attivazione di 150 classi di tempo pieno nelle scuole primarie di Milano e provincia. In proposito, la Direzione scolastica regionale per la Lombardia ha fornito le seguenti precisazioni sui vari punti evidenziati nell'atto di sindacato ispettivo. che il decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2009 non ha ridotto l'opzione del tempo scuola alle famiglie a due sole soluzioni, tempo normale-tempo pieno, ma all'articolo 4, comma 3, ha previsto nel tempo normale differenti articolazioni dell'orario settimanale, più precisamente 24, 27 fino a 30 ore, contemplando inoltre il modello delle 40 ore corrispondenti al tempo pieno. Si è così ampliata rispetto al passato la possibilità di scelta delle famiglie. L'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia ha tempestivamente predisposto le dotazioni organiche sulla base dello schema di decreto interministeriale trasmesso in allegato alla citata circolare n. 37 del 13 aprile 2010, poiché l'attesa della formalizzazione dello stesso avrebbe compromesso tutte le operazioni connesse alla mobilità territoriale e professionale dei docenti, che necessitano di una determinata tempistica per assicurare il regolare avvio dell'anno scolastico. Comunque, tutte le determinazioni assunte avranno effetto a partire dal 1° settembre 2010. In provincia di Milano, ove da parte delle famiglie è prevalsa l'opzione del tempo pieno, sono state autorizzate per la scuola primaria, nella previsione per l'anno scolastico 2010-2011, lo stesso numero di classi a tempo pieno autorizzate nel precedente anno scolastico, così come previsto dal suddetto L'affermazione che la provincia di Milano è al di sotto della media regionale del rapporto insegnanti-studenti deve intendersi nel senso che in essa ogni insegnante ha meno studenti di quanti ne abbia un insegnante di altra provincia, quindi tale rapporto è più favorevole rispetto alle altre.

in tutte le classi a tempo pieno sono garantite le 40 ore settimanali comprensive dell'insegnamento frontale (30 ore) e le 10 ore per la mensa. Tenuto conto che l'orario di due insegnanti per classe è complessivamente di 44 ore (ogni insegnante ha per contratto 22 ore di insegnamento frontale più 2 ore di programmazione di programmazione settimanali), ogni classe di tempo pieno comporta l'attribuzione di 4 ore in più di docenza rispetto all'esigenza delle 40 ore settimanali. Su tali ore in più, che costituiscono le cosiddette compresenze, si è operata una riduzione che è stata diversificata nelle varie istituzioni scolastiche. Complessivamente, in tutte le classi a tempo pieno si è assicurata una dotazione organica di 41 ore (un'ora in più rispetto alle 40 previste dal tempo scuola). La riduzione da 44 ore a 41 sulle compresenze comporta una conseguente riduzione dei posti, che è stata attuata gradualmente tenuto conto delle dimensioni delle istituzioni scolastiche, per cui in quelle con dimensioni minori (fino a 30 posti) si è ridotto un solo posto anziché due, fino ad una riduzione massima di 4 posti solo nelle scuole con organico superiore a 70. Con tali accorgimenti, in alcune scuole il monte ore assegnato per il tempo pieno è salito da 41 a 42 ore. Come può evincersi da quanto sopra, l'esigenza dell'utenza rispetto alle 40 ore settimanali è stata soddisfatta e sono state attribuite per ogni classe disponibilità in più da utilizzare nell'organico d'istituto,

delle situazioni di squilibrio a livello regionale nel rapporto insegnanti-alunni, che vedevano sfavorite altre realtà provinciali, ove l'offerta del tempo pieno non è così sviluppata, pur a fronte di richieste delle famiglie. Quanto operato non compromette affatto la promozione di un piano di sviluppo triennale d'intesa con le Regioni e gli enti locali, ma anzi è in linea con le indicazioni affinché tutte le maggiori economie che si verificheranno dovranno essere impegnate nel modello di estensione del tempo pieno.

quel capitolo e incominciamo a parlare di quello che sta facendo questo Governo. Per la parte che corrisponde non alla relazione introduttiva, ma al quesito vero e proprio, relativo alle classi a tempo pieno, per alcuni aspetti potrei potrei dichiararmi soddisfatta, nel senso che il Governo ha risposto alle domande che erano state poste. Ne deduciamo

per lo sviluppo del tempo pieno, oggi lo scarto tra la domanda e l'offerta, che è quello che interessa,

le richieste di tutti. E il Governo sta raccogliendo quello che ha seminato perché, avendo fatto la scelta del maestro unico e delle 24 ore, così reclamizzata, ed avendo abolito il modello più diffuso, che in Italia non era il tempo pieno (a Milano

Ora, lei stesso mi parla delle 4 ore residue; 4 ore residue vuol dire che il tempo pieno che si sta preparando per i nostri bambini è basato sulle 24 ore del famoso maestro unico, su cui vien fatto l'organico,

Quindi, dopo averci teorizzato, caro Sottosegretario, che il maestro unico era importante, perché i bambini avevano bisogno di un'unica figura educativa

l'anno scorso. Per il prossimo anno scolastico le scuole sono al buio e quindi non sono in grado di fare la previsione: altro che i criteri di previsione! Quindi, o siamo di fronte a una specie di congiura di massa, in cui tutti (dirigenti, insegnanti, genitori) congiurano contro il Governo e dicono menzogne, chiedendo i soldi ai genitori per riuscire a garantire l'ordinaria gestione della scuola

La Gelmini adesso ha avuto un figlio. Aspettiamo che cresca un po', così magari capirà che un'insegnante normodotata, con 26-27 bambini (perché adesso siamo a questi numeri) di numeri) di 7-8 anni, non li può portare in laboratorio tutti insieme. Ci proverà la Gelmini e vedremo. Chiunque, non dico abbia esperienze pedagogico-didattiche, ma abbia tirato su tre figli, sa che non si può, per ragioni di sicurezza, ma soprattutto per ragioni di apprendimento. Quindi, questa teorizzazione secondo cui le copresenze sono uno spreco,

Signor Presidente, è noto agli onorevoli interroganti che la scuola in ospedale da evento episodico, legato alla sensibilità di operatori e di istituzioni, si è trasformata in una struttura scolastica reale reale ed organizzata nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa delle scuole autonome. L'assegnazione di risorse derivanti dalla legge n. 440 del 1997 che ha istituito il fondo per l'arricchimento l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, garantisce il funzionamento delle sezioni ospedaliere e l'attivazione di progetti di istruzione domiciliare per ciascuna Regione. La risposta dell'Amministrazione per queste situazioni è finalizzata a garantire sempre il diritto allo studio e alla formazione della persona, anche in situazioni di difficoltà. È importante anche in questa sede sottolineare il ruolo significativo che svolge il docente in ospedale. Egli, infatti, oltre a garantire un ponte tra la famiglia e l'ospedale, tra la scuola e il mondo, ha anche il delicato compito di promuovere il diritto all'istruzione in un contesto così delicato e complesso. L'attività didattica, rivolta ai bambini e agli adolescenti ricoverati nelle strutture ospedaliere, o seguiti in regime di *day hospital* o di istruzione domiciliare, riveste un ruolo rilevante, in quanto garantisce agli stessi il diritto all'istruzione e al recupero del loro equilibrio psico-fisico, oltre a dare un contributo decisivo al recupero della dispersione scolastica dovuta alla malattia. Come già noto, la direttiva del Ministro n. 93 del 2009, concernente l'individuazione degli interventi prioritari e criteri generali per la ripartizione delle somme, per le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi stessi, ai sensi dell'articolo 2 della legge del 1997, ha previsto per l'anno 2009 iniziative finalizzate al potenziamento e alla qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni ricoverati in ospedale o seguiti in regime di *day hospital*. Anche quest'anno l'ammontare delle risorse assegnate per tali finalità, 3 milioni di euro, testimonia l'attenzione dell'Amministrazione per questa peculiare offerta formativa che si sviluppa in contesti di notevole complessità, sia che si tratti di sezioni ospedaliere, sia del domicilio degli studenti temporaneamente malati. La direttiva è stata registrata alla Corte dei conti in data 14 gennaio 2010 e a seguito della registrazione il Ministero ha richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze il provvedimento di variazione di bilancio, che è in corso di emanazione. Nel contempo il Ministero, con apposita circolare, ha già proceduto a dare comunicazione agli Uffici scolastici regionali dell'ammontare delle risorse finanziarie stanziate per la scuola in ospedale e per l'istruzione domiciliare per l'anno scolastico 2009-2010 ed a trasmettere il piano di riparto delle risorse attribuite, a seguito del monitoraggio delle attività, a ciascun Ufficio scolastico regionale. Gli Uffici scolastici regionali, sulla base della suddetta circolare, hanno provveduto ad approvare definitivamente e a realizzare i progetti di istruzione domiciliare, gli unici rimasti in sospeso, in attesa della certezza delle risorse. Alla data attuale risulta che tutti gli interventi sono in corso e che non vi sono, in nessun territorio, situazioni di interruzione degli interventi connessi a questa fascia di alunni, sia in ospedale che a domicilio.

cofirmataria. Questa interrogazione è nata in seguito a una serie di preoccupazioni che sono state poste proprio riguardo alla possibilità di dare corso a queste attività di studio per i bambini e le bambine malati molto gravi, purtroppo,

Lei ha fatto cenno alla legge n. 440 del 1997, al fatto che i 3 milioni di euro che dovevano essere stanziati per la scuola in ospedale e a domicilio sono stati finalmente stanziati e questo è un fatto positivo, però, faccio notare che questo avviene quando ormai siamo a fine anno scolastico e quindi per gli Uffici scolastici regionali è stato sicuramente difficile poter disporre in precedenza della possibilità di dare esito alle molte richieste che sono state fatte proprio in ragione della mancanza di certezza riguardo alla disponibilità Ecco, io vorrei attrarre l'attenzione sul fatto che dietro a questa disattenzione c'è probabilmente anche un fatto culturale: nonostante da molti anni ci sia una Convenzione dei diritti internazionali per l'infanzia, i bambini sembrano ancora privi di fatto di questi diritti soggettivi. diritti soggettivi. Chi è della mia generazione ricorda che, ad esempio, si pensava che i bambini non soffrissero. Chi di noi non si ricorda di aver sopportato operazioni di adenoidi o di tonsille senza essere sedati? Oggi questo sarebbe improponibile. Poi si è acquisito che culturalmente i bambini soffrono e che il dolore va eliminato. Poi si è capito che per i bambini è un trauma stare in ospedale perché questo dà l'idea di essere abbandonati dai propri genitori, è fonte di dolore, quindi si è capito che bisognava lasciare i genitori vicino ai propri bambini anche durante il ricovero. Poi si è operato per una riduzione dei tempi di ricovero e non solo per ridurre i costi della sanità, ma per rendere appunto possibile al bambino anche malato gravemente di condurre una vita il più possibile normale e si è capito che ridurre i tempi di ricovero poteva facilitare la guarigione. Oltretutto, si è pensato che fosse importante migliorare la qualità della vita: e l'ambito familiare è sicuramente il luogo migliore dove il bambino può essere curato. si è pensato che la scuola in ospedale o a domicilio fosse uno strumento indispensabile all'interno appunto di questo progetto di qualità della vita anche per per i bambini malati, perché fa sentire i bambini meno malati, perché li rende più uguali ai loro coetanei, perché dà loro la possibilità di esercitare un diritto che è costituzionale, quale quello all'istruzione. Vorrei ricordare che quest'attività scolastica, sia all'interno degli ospedali che a domicilio, viene fatta da molto tempo da insegnanti preparati perché vengono attivati dei corsi di formazione specifici per questi insegnanti, proprio perché questi corsi rientrano di fatto a pieno titolo nel programma terapeutico del bambino interessato. Di fronte a questo io credo che noi dobbiamo essere preoccupati del fatto che la questione si ripresenti il prossimo anno. Da qui la mia parziale preoccupazione. I fondi sono stati dati ora che siamo alla che siamo alla fine dell'anno scolastico 2009-2010. Come si presenterà la situazione ad ottobre per l'anno scolastico 2010-2011 se non abbiamo certezza che si opererà per tempo in modo che tutti i bambini che lo richiedano possano frequentare questi corsi?

e con la certezza dei fondi che sono necessari a disposizione secondo anche quanto prevede la legge.

L'organico magistratuale del tribunale, di cui fanno parte tabellarmente il capo dell'ufficio e nove giudici togati, presenta, allo stato, una sola vacanza nelle predette nove unità di giudice. Faccio presente, inoltre, che con delibera del Consiglio superiore della magistratura del 14 gennaio 2010 è stata individuata la figura del presidente del tribunale nella persona del dottor Michele Cristino il quale, in data 25 marzo 2010, ha preso possesso dell'ufficio. Segnalo, poi, che presso il predetto ufficio sono attualmente in servizio anche quattro unità di giudice onorario di tribunale. Ad ogni buon conto, tengo ad evidenziare, sul piano generale, che per far fronte alla situazione di scopertura degli uffici giudiziari meno richiesti, il Governo ha recentemente emanato il decreto-legge n. 193 del 2009, convertito nella legge n. 24 del 2010, recante, tra le altre, diverse norme in materia di trasferimento d'ufficio dei magistrati nelle sedi disagiate. In attesa della piena operatività delle complesse modifiche introdotte all'ordinamento giudiziario è stata altresì prevista l'adozione di urgenza di alcune misure contenute nel disegno di legge di iniziativa governativa Atto Senato n. 1440. Tra queste, quella che consente al Consiglio superiore della magistratura, nei casi in cui difettino aspiranti al trasferimento presso le sedi disagiate, di procedere, fino al 31 dicembre 2014, al trasferimento d'ufficio non solo dei magistrati cosiddetti ultradecennali, ma anche di quelli che abbiano conseguito la prima o la seconda valutazione di professionalità. Quanto alle principali novità normativamente introdotte, è stato previsto un ampliamento del numero delle sedi annualmente individuabili come disagiate da parte del Consiglio superiore della magistratura (che potranno quindi arrivare sino ad ottanta), nonché dei magistrati ivi destinabili (che potranno giungere fino a Oltre a ciò, è stata introdotta la cosiddetta assegnazione provvisoria di sede, che consentirà di coprire le sedi meno ambite, anche attraverso il sistematico utilizzo dei magistrati di nuova nomina. Tra gli ulteriori strumenti forniti dal Governo al Consiglio superiore della magistratura nella qualità di organo deputato alla copertura di organico delle sedi, ivi comprese quelle disagiate, segnalo, inoltre, il previsto rafforzamento dello strumento strumento del trasferimento d'ufficio, in deroga ai divieti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 160 del 2006 e la possibile attribuzione ai magistrati nominati con decreto ministeriale 2 ottobre 2009 delle funzioni requirenti al termine del loro tirocinio, nel caso in cui, alla data di assegnazione delle sedi, sussista una scopertura di organico superiore al 30 per cento in relazione ai posti per cui è consentito il trasferimento d'ufficio. Oltre a ciò, evidenzio che, per effetto della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il ruolo organico della magistratura è stato ulteriormente ampliato in ragione di quarantadue unità e che le stesse verranno distribuite tra gli uffici giudiziari secondo criteri improntati a realizzare un riequilibrio dei carichi di lavoro e sulla scorta dei valori medi rilevati con riferimento ai procedimenti sopravvenuti per unità di magistrato in organico. In tale contesto, saranno tenute in debita considerazione le esigenze di incremento dell'ufficio in questione, fermo restando le imprescindibili valutazioni comparative.

Le vacanze nell'organico amministrativo sono, quindi, contenute in numero di quattro unità ed interessano una la figura del direttore di cancelleria C3, una quella di cancelliere C2, una quella di ausiliario B1 e una quella di operatore giudiziario B1. La scopertura esistente nell'ufficio si attesta, pertanto, nella misura dell'11,43 per cento. Allo stato, infatti, risultano coperti gli organici di cancelliere C1 e B3, così come risulta coperto anche l'organico di operatore giudiziario B2, di autista e di un ausiliario A1. Detto ciò, pur senza sottacere le difficoltà comunque connesse alla pur esigua scopertura di personale del suddetto ufficio, non si può non valorizzare il ruolo che spetta al capo di corte per la risoluzione nel breve periodo di tali problematiche. Nello specifico, mi riferisco alle applicazioni di personale da altri uffici del distretto ad opera del presidente della corte di appello, nei modi previsti dall'articolo 14 dell'accordo sulla mobilità interna del 27 marzo 2007, ovvero ai comandi di personale da altre Amministrazioni. Si tratta, infatti, di interventi più celeri, attraverso i quali compatibilmente con le esigenze di servizio degli altri uffici giudiziari del distretto è possibile acquisire temporaneamente personale per fronteggiare situazioni di disagio.

presso il tribunale di Melfi, che ha una dotazione di dieci magistrati, ben due di loro erano stati trasferiti, due erano in astensione per gravidanza, altri due avevano presentato domanda di trasferimento e due uditori giudiziari erano al lavoro, ma, come sappiamo, non potevano essere dediti all'esercizio di funzioni monocratiche. Quindi, si appalesava un rischio di totale paralisi di quel tribunale e fu, come dire, questa ragione un po' eccezionale, questo timore, che spinse me e i colleghi a sollecitare un intervento e un provvedimento del Ministero, che è avvenuto perché ben quattro nuovi magistrati sono stati assegnati. Per questa ragione mi sento di esprimere una soddisfazione per l'attenzione che il Ministero ha dedicato. Si tratta di un'area, quella della Basilicata, dove in genere la funzione della magistratura ha protetto ha protetto abbastanza la Regione dalla infiltrazione e anche dallo strutturarsi di organizzazioni criminali. Il lavoro della magistratura è stato significativo, soprattutto nell'area di Melfi, dove vi è stata negli ultimi anni una recrudescenza di attività criminali. Restano preoccupazioni, signor Sottosegretario, che lei stesso ha citato in ordine a due domande di trasferimento che potrebbero concretizzarsi nel mese di settembre di due magistrati (scenderemmo di nuovo a sette unità). C'è poi un punto di criticità, che ho visto presente nella sua risposta, che riguarda le figure di cancelliere e la mancanza di un dirigente di cancelleria, di una figura apicale, che pure pesa sull'ordinaria attività di quel tribunale. L'avevo appunto compresa questa deficienza nelle sue considerazioni, me ne compiaccio e e sono convinto che il Governo e il Ministero faranno di tutto per evitare che una crisi scongiurata che ha riguardato i magistrati possa essere invece determinata dall'assenza di un numero così cospicuo di cancellieri.

affinché la risposta ai quesiti sollevati dal senatore Di Giovan Paolo possa risultare chiara, è necessario operare alcuni distinguo e separare tra le situazioni segnalate quelle apparentemente già concluse da quelle in via di definizione. Un primo imprescindibile chiarimento riguarda, invero, la riutilizzazione delle case mandamentali soppresse. Molte delle strutture indicate dal senatore interrogante sono, infatti, case mandamentali che, nella maggior parte dei casi, non sono più nella disponibilità di questa Amministrazione. Si tratta di strutture che, a causa della loro originaria destinazione, presentano notevoli carenze sia per le dimensioni decisamente ridotte, sia per l'assenza di sistemi di sicurezza adeguati, oltre che per la mancanza di spazi alloggiativi per il personale e di spazi trattamentali per i detenuti. La loro attivazione,

sono state soppresse, in un arco temporale compreso tra il 1991 ed il 2009, mentre le relative strutture sono state restituite ai rispettivi Comuni, in quanto pertinenza del patrimonio comunale. La casa circondariale di Pinerolo è stata definitivamente chiusa nel 1998, atteso che le precarie condizioni igienico-sanitarie e le caratteristiche strutturali del manufatto (non funzionante perché incompleta), sarà cura di questa Amministrazione provvedere, a breve, ad una disamina approfondita delle loro condizioni, verificando nel concreto la convenienza di un loro mantenimento, stante il basso indice di sicurezza delle strutture attualmente in uso.

È questo il caso del penitenziario di Reggio Calabria, Arghillà, che risulta ancora in fase di realizzazione. La costruzione del nuovo istituto - di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - è stata, infatti, interessata da un lungo contenzioso, che ha dilatato i tempi relativi al completamento dell'opera.

La competente direzione generale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha, pertanto, provveduto tempestivamente alla revisione del progetto, inviando, in data 16 dicembre 2009, copia degli elaborati al suddetto provveditore, il quale, a sua volta, ha assicurato la rapida elaborazione del progetto esecutivo di completamento generale Per completezza di informativa, rappresento che la struttura già edificata è composta da un padiglione detentivo da 150 posti, matricola e servizi detentivi; sono, invece, ancora da realizzare un padiglione detentivo da 100 posti, l'allacciamento delle fognature, la strada di accesso all'istituto, la caserma agenti, gli uffici e gli alloggi. Analogo discorso vale per l'istituto Barcaglione di Ancona, che risulta attualmente in fase di ultimazione. Premesso che la parte già funzionante dell'istituto consente di poter ospitare 24 detenuti, rappresento

per l'esecuzione di tutte le opere minimali necessarie alla completa attivazione dell'istituto. All'esito di tali lavori, saranno, quindi, disponibili ulteriori 134 posti. In estrema sintesi, l'istituto penitenziario, una volta completata l'attivazione, consentirà di ospitare 182 detenuti.

Orbene, chiarite le situazioni segnalate, ricordo a tutti che è stato recentemente approvato dal Consiglio dei ministri, e sta per essere trasmesso alle Camere, un complesso di interventi normativi, noto come "Piano carceri", che poggia su quattro pilastri. si prevede la proclamazione dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2010 per consentire una rapida edificazione dei nuovi edifici carcerari. La procedura di emergenza, che seguirà lo stesso schema usato

Nell'ambito degli interventi governativi finalizzati ad una celere e fattiva risoluzione delle problematiche presenti in ambito carcerario, si segnala il disegno di legge n. (Atto Camera), d'iniziativa del ministro Alfano. Tale disegno contiene diverse misure dirette ad attenuare la tensione detentiva collegata alla elevatissima percentuale di detenuti

ovvero di centri religiosi e che, pertanto, si tratta di una forma di detenzione ampiamente sperimentata e che ha prodotto buoni risultati. Naturalmente, la regola generale affermata nell'articolo 1,

dall'ordinamento penitenziario, in modo da garantire decisioni certe e rapide. In particolare, il provvedimento è emesso da un giudice monocratico - il magistrato di sorveglianza - sulla base di un'istruttoria cartolare ed un contraddittorio differito. I casi in cui non può essere prevista la detenzione presso il domicilio sono tassativamente indicati. Giova evidenziare, infine,

Vale da ultimo evidenziare che il disegno di legge contiene anche alcune disposizioni per i condannati che versano in condizioni di tossicodipendenza. Il comma 7 dell'articolo 1 del suddetto disegno di legge - così come riformulato dall'emendamento 1.500 del Governo - prevede che per i condannati sottoposti

grande soddisfazione per il fatto che partecipa ai lavori (lo voglio dire pubblicamente), molto spesso dà un contributo concreto e fa onore al ruolo del sindacato ispettivo, nel senso che ho ricevuto più risposte di quelle che avevo richiesto. Per quanto Per quanto riguarda le situazioni che segnalavo di alcuni istituti carcerari, alcuni in condizioni di cui non si conosceva lo stato dell'arte, abbiamo ricevuto risposta e su questo c'è sicuramente un chiarimento (andrebbe fatto continuamente, d'abitudine); di alcune

12 punti sui quali il prossimo anno saremo tutti insieme chiamati a ragionare e a rendere conto. Si va in questa direzione: alcune parti del Piano carceri e l'attenzione che si pone sulla materia È anche l'idea che noi abbiamo, cioè che si riparta dallo spirito della legge Gozzini e, ormai lontani due anni e mezzo dalle elezioni, non ci sia più bisogno di sollevare lo spauracchio della sicurezza, quanto invece di porsi il problema che vi sono quasi 30.000 unità

ovviamente concordiamo sul fatto che, qualora vi fosse un'autorità nazionale per i diritti umani (su cui si sta lavorando e a cui il sottosegretario Scotti, tra l'altro, ha dato riscontro),